scopriamo, leggendo un po' meglio le carte (anche se nelle poche ore che il Senato ha avuto a disposizione per poterle esaminare), che Equitalia non cambia affatto: cambia solo la targa all'esterno dei palazzi dove ha sede. Doveva, peraltro, essere il decreto-legge che, partendo da Equitalia, avanzava sul terreno di quel fisco amico, obiettivo di tanti quasi sempre fallito. infatti, invece di andare verso il fisco amico o quella *tax compliance* - come si dice oggi - ci si mette sotto i piedi anche quel poco che resta di un codice del contribuente sempre disatteso ad ogni decreto-legge economico e fiscale. Doveva essere una semplificazione e invece solo i nuovi adempimenti, che riempiono tre pagine scritte fitte fitte,

Se hanno protestato i commercialisti, signora Presidente, figuriamoci quanto protesteranno i contribuenti quando scopriranno che, dall'accertamento alla riscossione, in un'unica soluzione, un unico mostro entrerà nella loro vita, potendo utilizzare quelle importanti e delicate banche dati non solo ai fini della riscossione ma chissà a quali altri. È un tema assai delicato quello che viene affrontato in questo decreto-legge, disattendendo, da parte del Governo, ogni logica verso un fisco moderno e un sistema di controllo di lotta all'evasione che deve operare nelle forme più severe possibili, ma non può impedire alle persone di essere titolari della loro vita, del loro contratto di lavoro, della loro contribuzione previdenziale, di tutto ciò che pagano e versano, che deve servire a sostenere le esigenze di una vita lavorativa e poi pensionistica; al contrario, in questo decreto viene utilizzato ai fini del pagamento delle tasse. Ma per il Governo, che avrebbe l'ambizione di ridurre la pressione fiscale, questa è forse la più tragica occasione mancata. Persino alla vigilia di una consultazione elettorale così importante non viene in mente al Governo e alla sua maggioranza che il principale oggetto della nostra attenzione e tutela deve essere proprio il cittadino italiano, il contribuente italiano, pur nell'ambito di una giusta quanto corretta lotta all'evasione fiscale. Ma si capisce poi presto perché non poteva che essere così: con la scusa di cambiare nome a Equitalia, in realtà, attraverso un decreto-legge fiscale si immagina nuovo gettito erariale,

Quindi è un decreto che serviva a coprire, a fare cassa e, se serve a fare cassa, vuol dire che dal cambio del nome di Equitalia gli italiani avranno solo da rimetterci.

che la Ragioneria quota risultanti dai pignoramenti che saranno immediatamente esecutivi quando entrerà in vigore, tra qualche giorno, la procedura; e con i pignoramenti dei beni degli italiani noi dobbiamo andare a coprire le spese che sosteniamo per l'ondata migratoria che nel nostro Paese non si arresta. E non si arresterà perché questo Governo, che è forte con i contribuenti italiani e debole invece con gli europei, con gli altri Paesi e, soprattutto, con l'Unione europea,

altro importante. Il funzionario che guiderà tutta l'attività di controllo sugli *hotspot* europei, soprattutto quelli italiani, sarà un inglese nell'epoca della Brexit, se gli inglesi riescono a essere più valutati e considerati degli italiani su un tema come quello dell'immigrazione, vuol dire che noi siamo davvero messi molto male, peggio della Brexit. E questo Governo riuscirà con la sua azione debolissima e incapace in Europa a deludere ancora una volta le attese di tanti italiani che pensano che, con un solo si potrebbe davvero cambiare la situazione del nostro Paese. Servirà invece un grande «no» per fermare un Governo che l'unica cosa che sa fare è studiare un decreto fiscale, ingannando gli italiani che produrrà nuovo gettito di tasse allo Stato il quale dovrà coprire sempre maggiori spese per un'immigrazione che non controlla, non governa e che decidono altri. La decidono persino quelli che dall'Europa hanno deciso di uscire. allora, signora Presidente, che sia arrivato il momento delle parole e della verità. Da qui ai prossimi quindici

Questo decreto è un esempio del modo di governare di Renzi, del modo di ingannare i cittadini: un decreto-legge approvato in trentuno giorni tra Camera e Senato con voto finale di fiducia; decreto che parla di scioglimento di Equitalia, di semplificazioni, di finanziamenti per esigenze indifferibili: falsità, menzogne. Equitalia non verrà abolita, ma verrà istituita al suo posto l'Agenzia delle entrate-riscossione. Si tratta solo di un cambio di nome e di forma giuridica. Il nuovo statuto sarà approvato dal Governo. La nuova Agenzia avrà il controllo diretto da parte del Governo, diventerà un braccio operativo del Governo sul fronte fiscale. L'articolo 3 prevede che la nuova società di riscossione potrà controllare l'ammontare del conto di ogni contribuente, l'ammontare dello stipendio e della pensione; potrà fare una radiografia completa e preventiva dello stato patrimoniale di ogni cittadino italiano. Si promuove, quindi, il potenziamento della riscossione per rendere più efficace il pignoramento di stipendi, salari e indennità. Altro che fisco amico, come ci è stato raccontato da Renzi: falsità, menzogne. L'articolo 4 prevede nuove disposizioni per il recupero dell'evasione e, in particolare, nuovi adempimenti per le partite IVA: comunicazioni analitiche di tutte le fatture emesse e ricevute comunicazioni trimestrali dell'IVA. Altro che semplificazione: renderete un inferno la vita dei cittadini, dei contribuenti, delle famiglie. Avete provocato persino la protesta dei commercialisti. I nuovi adempimenti diventeranno nuovi costi per i cittadini. Otto nuovi adempimenti fiscali e sanzioni spropositate: un mero errore formale di un euro produrrà una sanzione minima di 5.000 euro. Non lo diciamo noi: lo dice l'associazione dei commercialisti, che sono scandalizzati dalle norme di questo decreto. La moratoria delle cartelle esattoriali: niente sanzioni e more se si paga in fretta. altro grande inganno. Chi potrà avvalersi di tale opportunità se dovrà versare il 70 per cento delle somme dovute al fisco entro la fine 2017 e il restante 30 per cento nel 2018? Solo chi gestisce grandi capitali, cioè i grandi evasori, chi potrà indebitarsi con le banche, e non certamente i comuni cittadini o le piccole imprese, che non riescono nemmeno a pagare le tasse anno per anno. Volete solo far cassa nel 2017. Avete bisogno di denaro fresco da spendere per costruire il vostro consenso. Ma non vi saranno le entrate che vi aspettate, come non ci saranno dalla *voluntary disclosure*. Approvate questo decreto-legge per inserire nella legge di bilancio e di stabilità entrate fasulle pur di far stare in piedi le vostre spese elettoralistiche. E poi ci sono gli ultimi articoli, che nulla hanno a che fare con un decreto fiscale e con investimenti indifferibili e urgenti. Si tratta esclusivamente di mance referendarie, di elargizioni a pioggia per portare consensi alla campagna governativa per il "sì". Ne cito solo alcune: 600 milioni ai Comuni che collaborano con il Governo alla creazione di centri d'accoglienza dei migranti; premi senza logica, senza giustizia. Ogni Comune ha diritto ad una distribuzione equa delle risorse, a prescindere dal fatto che aiuti o no Renzi e Alfano nella folle politica dell'invasione. E poi ci sono 600 milioni alla Regione Campania di De Luca, per pagare i debiti contratti con la società di trasporto ferroviaria regionale; e altri 90 milioni alla Regione Molise, per i debiti contratti con Trenitalia. La solita logica: chi spende male i soldi pubblici viene premiato; chi li spende bene viene preso in giro. Di più: chi fa campagna referendaria per Renzi ottiene investimenti pubblici dal Governo, gli altri no.

a partire dalla buona scuola. Con questo decreto-legge, approvato tra Camera e Senato in soli trentuno giorni con la fiducia, dimostrate che il Governo non ha bisogno di poteri speciali per approvare le leggi e che il bicameralismo non è un problema, ma è un alibi. Già ora usate e abusate della Costituzione per fare ciò che volete. Chissà poi, se venisse approvata la vostra riforma, cosa accadrebbe in queste Aule. La verità è che Renzi vuole togliere potere alle autonomie locali e ai cittadini per fare ciò che vuole, senza nemmeno chiedere il permesso. Se oggi il cittadino ha la sensazione di contare poco nelle decisioni politiche, un domani, se passerà la riforma, questa sensazione diventerà una certezza. I cittadini non eleggeranno più i propri rappresentanti, ma questi verranno nominati da altri politici nei consigli regionali; stesso metodo della nomina dei consiglieri e presidenti delle Province. Quello che volete mettere in atto è il superamento della democrazia: sottrarre sovranità popolare ai cittadini, perché i poteri a cui Renzi risponde hanno terrore della democrazia. La variabile del voto popolare nella realizzazione dei loro progetti è una variabile che temono, essere ridimensionata, eliminata, e Renzi ha varato una riforma per raggiungere questo obiettivo. Renzi punta a ottenere uno sbandierato,

e non aderiscano al modello Renzi-De Luca del voto di scambio. Il diritto di voto non deve essere svenduto a Renzi e a nessuno ma, deve perché non ha prezzo. La Lega Nord vota no a questo decreto-legge; vota no alla fiducia al Governo Renzi; voterà no il 4 dicembre a una riforma che non è nell'interesse dei cittadini, ma è nell'interesse del palazzo. Noi diciamo no.

avevamo avuto un approccio nei confronti del decreto fiscale di grande interesse e volontà di partecipazione alla modifica di quello che riteniamo essere uno dei punti deboli del nostro sistema statuale. La pressione fiscale eccessiva, ma anche le forme di esecuzione per la riscossione delle tasse sono uno degli aspetti che riteniamo più scandalosi del nostro sistema Paese. la dichiarata volontà di eliminare Equitalia si sposava, nel nostro sentire, con la volontà di dare ai contribuenti italiani un sistema di riscossione più equo, davvero un sistema in cui il fisco non sia visto, nell'immaginario collettivo, come il satrapo impositore che persegue il cittadino contribuente, ma come lo coadiuva, lo aiuta nell'esercizio doveroso del pagamento delle tasse dovute. Invece ci troviamo di fronte a un'operazione di facciata, un'operazione di facciata, che ha bisogno del voto di fiducia per consentire, ancora una volta, che non vi sia un libero dibattito che possa portare miglioramento a un provvedimento di legge che non si capisce a chi vuole portare giovamento:

che ormai si avvicendano l'uno dopo l'altro, non hanno più la capacità, la potestà, la possibilità di far fronte anche al dovuto nei confronti del fisco. Ebbene, questo provvedimento, la cosiddetta

Non esiste piccola o media impresa che possa aderire a una rottamazione che prevede l'immediato pagamento, nell'esercizio 2017, del 70 per cento della somma dovuta. Un'operazione di questo genere non porta giovamento neanche alle tasche dello Stato. Infatti voi, con questo provvedimento, avete introdotto una una manovra che avreste considerato scandalosa se solo fosse stata messa in campo da un Governo di altro segno, da un Governo di centrodestra. Voi introducete un condono

quindi, non porterà benefici neanche alle tasche dello Stato per l'impossibilità di adesione a una rottamazione così congegnata.

fiscale, in cui si prevede una rottamazione agevolata per i petrolieri, per le aziende che operano nel settore del gas e degli idrocarburi: per loro viene prevista una rottamazione diversa;

residua dei pagamenti delle loro cartelle. Si ha così un doppio metro, una doppia corsia: una corsia larga, comoda e veloce,

perché avete voluto fare un'ennesima operazione di facciata con il sistema radiotelevisivo, che è quello di Stato ed è pagato con soldi dei contribuenti, che fa un'operazione assolutamente incredibile di imbonimento. imbonimento. Negli ultimi giorni si continua a ripetere che si è aggiustato al rialzo l'andamento del PIL allo 0,8

quindi l'aggiustamento sarà in positivo rispetto all'ultimo trimestre, ma è in assoluto negativo rispetto alle previsioni fatte dal Governo all'inizio dell'anno.

e l'indebitamento ulteriore, a firma Renzi, in questo Paese è già di 112 miliardi rispetto alla precedente gestione. È un indebitamento che continua. Che fine hanno fatto, allora, le dichiarazioni per cui erano delinquenziali le politiche precedenti che avevano consegnato alle future generazioni un debito colossale? un debito colossale? Voi lo state soltanto aumentando. Il nostro debito pubblico non solo non diminuisce, ma aumenta di altri 112 miliardi. Come pensate voi alle generazioni future? In quale Paese immaginate che possano vivere le nostre nuove generazioni, ulteriormente appesantite dall'azione di debito? Non pensiate - ve lo dico il cuore in mano - che possano essere i cosiddetti poteri forti, la grande finanza internazionale a salvare questo Paese. Il nostro Paese, con le sue capacità, con la forza che deriva dalla sua struttura di impresa, piccola e media,

pignoramenti di aziende e case. Vedremo ancora - lo temo - atti di autolesionismo da parte di chi non si vuole rassegnare; quando si vede togliere la propria casa o si vedono porre i sigilli alla propria azienda,

perdere di competitività e capacità economica a causa di un sistema che uccide le piccole e medie imprese. E in questo sistema rientra anche quello fiscale, quello del settore bancario e dell'accesso al credito. Ebbene, contro questo sistema, non solo il Governo non dà alcuna arma e alcuna possibilità di lotta, ma addirittura ci si associa. Questo è un Governo che avverte e sostiene le sensibilità che provengono dal mondo finanziario e bancario, dal mondo delle produzioni multinazionali, completamente sordo alle esigenze della nostra struttura imprenditoriale e ai richiami

provvedimento è parte integrante della manovra di fine anno. Ne rappresenta l'elemento essenziale, provvedendo al reperimento delle risorse finanziarie

pertanto prescindere da una valutazione più complessiva, anche se il collegamento con la manovra di fine anno ha un carattere ambivalente, attribuendo al provvedimento un carattere inevitabilmente provvisorio. È evidente, infatti, che dovremo tornare a riconsiderare alcune norme quando il quadro sarà meglio definito. Siamo infatti in attesa del definitivo responso della Commissione europea, che sarà reso noto - ahimè - solo dopo il 4 dicembre. Vedremo allora come si potrà ricomporre quella diversità di valutazioni che finora è stata solo annunciata. Al momento, sulla scorta di documenti ufficiali, si può solo misurare il perimetro della divergenza. Si tratta più o meno di cinque miliardi - come ieri il senatore Milo ha avuto modo di dire - ai quali si dovrà fare fronte, in tutto o in parte, secondo l'evoluzione del possibile negoziato. E ci auguriamo che il Presidente del Consiglio ce la faccia a negoziare bene. Ne deriva pertanto che la stessa legge di bilancio, che la Camera dei deputati si appresta a varare - sappiamo che la Commissione ha lavorato fino a tardi ieri notte - dovrà tener conto di questa variabile esogena. Il Senato dovrà riconsiderare il tutto alla luce della nostra prospettiva e lì forniremo il nostro contributo. Dichiaro già il voto favorevole del nostro Gruppo, ma con la legge di bilancio noi dovremo dovremo avere quelle risposte in termini di riconduzione positiva della manovra di bilancio nei binari giusti, come riteniamo opportuno e non per critica, ma per costruire insieme una legge di bilancio che serva a tutti quanti noi. Nel frattempo, tuttavia, non possiamo esimerci dall'effettuare una valutazione di un testo che presenta molte luci e alcune ombre: ombre che abbiamo cercato di diradare con i nostri emendamenti, sui quali insisteremo quando la manovra avrà assunto un carattere più definitivo. La prima osservazione riguarda i grandi numeri. La manovra, come noto, comporterà un aumento del *deficit* di 12 miliardi di euro, pari allo 0,7 per

si riferiscono al ventilato aumento dell'IVA e delle accise (problema scongiurato per il 2017, ma non per gli anni successivi), oneri il cui valore, sempre per il 2017, è pari a 15,1 miliardi Paragonando le due cifre si può facilmente dedurre che l'intera manovra prevista risulta insufficiente per coprire quel «pagherò fiscale», come lo ha definito il vice ministro Zanetti in un suo brillante intervento giornalistico,

se l'è data specchiandosi, perché questo *vulnus* è partito proprio da lui e da una sua invenzione infelice,

40 di quel decreto-legge prevedeva un taglio delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali e, ancora oggi, fa una certa impressione vedere quella quarantina di pagine che costituiscono l'allegato *c)* del provvedimento, una tabella in cui sono minuziosamente elencate le 1.000 voci che potrebbero garantire un aumento di prelievo fiscale. Già allora si pensava a un riordino dell'intera materia, ma, come nel caso della *spending review*, l'unica cosa che è cambiata sono gli uomini preposti a individuare la rotta del cambiamento.

a trovare il modo di tappare quei buchi. Questa valutazione di carattere più generale non può impedire una più attenta valutazione di merito. Ieri il senatore Milo ci ha parlato dell'articolo 5-*bis*

Anche in materia di diritti audiovisivi sportivi si poteva fare meglio. Il nostro Gruppo lo ha più volte detto. Sono, infatti, numerose le istanze che sono giunte al nostro Gruppo a sostegno dell'ottimo lavoro fatto nella Lega Pro, nel tentativo di modificare quanto previsto nel decreto. Le istanze evidenziano in maniera chiara le difficoltà e le preoccupazioni economiche della serie A, B, lega Pro e lega Basket.

Non è chiaro nel testo al nostro esame il destino dei centri di riscossione diversi da Equitalia: continueranno a operare oppure saranno tagliati fuori dalle provvidenze previste per i contribuenti? Quest'ultima eventualità comporterebbe la loro crisi inevitabile, con riflessi diretti e immediati su centinaia di lavoratori

I grandi numeri depongono a favore della manovra, quelli piccoli la contraddicono in molti punti qualificanti. Il Gruppo AL-A si farà carico di questo problema non risolto quando, chiarito il quadro economico e quello politico, si tratterà di discutere della legge di bilancio. In quella sede, lo annuncio fin da ora, ci batteremo affinché gli emendamenti che abbiamo presentato, ma non presi in considerazione per causa di forza maggiore, ritrovino l'attenzione che meritano. Oggi noi daremo fiducia al Governo. Domani, se le nostre proposte costruttive non venissero prese in considerazione, ci adegueremo e valuteremo un voto diverso da quello odierno.

ossia l'equità e la semplificazione del rapporto fra il sistema fiscale e il contribuente, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate e riscossione e l'effettiva e maggiore autonomia degli enti locali in merito alle scelte per la riscossione dei tributi locali. In termini generali, con il provvedimento in esame si prosegue nel rafforzare le opportunità di ravvedimento da parte dei contribuenti e il consolidamento delle procedure di composizione in luogo di possibili contenziosi. Fra i punti rilevanti del provvedimento concordiamo con la decisione del Governo di riaprire i termini relativi alla *voluntary disclosure*. La riapertura delle procedure e dei termini evidentemente non può che confermare le regole che hanno già disciplinato l'azione Si tratta di misure che hanno introdotto, e ora ribadiscono, sostanziali novità nel rapporto tra sistema tributario e contribuenti, ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni di evasione fiscale. Le disposizioni relative alla riapertura della *voluntary* *disclosure* rappresentano un'ulteriore opportunità affinché i contribuenti decidano di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco. In ordine alla *voluntary* *disclosure* ribadiamo, come già richiesto con un ordine del giorno alla Camera dei deputati accolto dal Governo, l'auspicio che nell'esame parlamentare della legge di bilancio venga chiarito che, in forza dello Statuto speciale

in ordine all'analogo problema della Valle d'Aosta. Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-Maie.

credo che ormai il Governo Renzi abbia battuto ogni *record* per quanto riguarda le questioni di fiducia, superando largamente tutti gli Esecutivi che lo hanno preceduto. Anche oggi ci troviamo quindi di fronte al solito copione, con un uso e un abuso della decretazione d'urgenza - su cui abbiamo già avuto modo di intervenire già ieri nella

si vede, quando interessa al Governo si procede sempre molto rapidamente alla faccia delle presunte lentezze legate al bicameralismo perfetto.

il Governo Renzi si muove in politica economica su due linee

di una ricetta che si è già dimostrata assolutamente sbagliata e certamente non sufficiente, cioè la manovra sul lato dell'offerta, con misure

Noi riteniamo sostanzialmente che queste due linee hanno prodotto non solo risultati assolutamente insufficienti, ma sul lato della strumentalità elettorale anche dei danni dal punto di vista dei saldi e dei conti. La nuova versione di quest'ultima fase è la polemica con la Commissione europea, ma non su

sulla discussione su alcuni margini di flessibilità (non da dedicare agli investimenti), e non certamente nella messa in discussione degli assi portanti della politica europea, che è stata assolutamente sbagliata.

Anche questo decreto - lo dobbiamo dire con molta chiarezza - presenta tutti i vizi che ho descritto,

perché pensiamo che bisognerebbe intervenire massicciamente sul lato della domanda e non dell'offerta, quindi con politiche di investimento. Qualcuno potrà

terremoto: occorrerebbero degli investimenti enormi per la messa in sicurezza del nostro territorio dal rischio idrogeologico e la messa in sicurezza degli edifici. Serve una politica energetica diversa, quindi una massiccia dose di politiche di investimenti sociali.

ha fatto credere che l'intervento su Equitalia fosse legato alla rottamazione di tutte le cartelle, lasciando immaginare all'opinione pubblica che l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora fosse contenuta anche nel superamento di Equitalia. Invece, sappiamo tutti che questa è una misura di carattere straordinario

ha già pagato tutto rispetto ad altri che invece non lo hanno fatto e che oggi ne avranno un evidente vantaggio. Tra le altre cose, in questo decreto non si chiarisce assolutamente neanche se ci sarà una proroga per il regime giuridico dei contribuenti che dichiarano uno stato di difficoltà. Insomma, non siamo assolutamente d'accordo nel merito, per non parlare della *voluntary disclosure*, che significa l'ennesimo condono. In questo modo non facciamo né un'operazione di giustizia né un'operazione che possa servire davvero a questo Paese. Per questo il nostro è è un no chiaro, un no nel merito, un no alla fiducia, l'ennesima, posta da questo Governo. colleghi, la legge di delega fiscale del 2014 e i successivi decreti attuativi hanno tracciato la strada. Il disegno ispiratore di questo decreto-legge, arricchito dal lavoro parlamentare, è sempre lo stesso: costruire finalmente un nuovo e inedito rapporto tra il contribuente italiano e l'erario; un rapporto di leale collaborazione fondato sul reciproco affidamento ciascuno nel rispettivo ruolo: uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela dell'interesse generale e nel contempo a contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale. È un disegno ambizioso che avrà bisogno di molta cura legislativa e anche di tempo. Area Popolare voterà favorevolmente al decreto-legge fiscale, in quanto il lavoro svolto dai Gruppi parlamentari è stato dettato da un principio di equità e da una concezione del fisco come strumento per incentivare l'iniziativa economica dei cittadini, e quindi lo sviluppo. La raccolta fiscale e la spesa pubblica assumono un'importanza economica cruciale per ogni comunità civile e politica; pertanto, l'obiettivo verso cui tendere è una finanza pubblica capace di proporsi come strumento di sviluppo Ma sopratutto, la finanza pubblica viene accettata e assimilata dal contribuente unicamente quando si orienta al bene comune e quando si attiene ad alcuni principi fondamentali: il pagamento delle imposte come specificazione del dovere di solidarietà, razionalità ed equità nell'impostazione dei tributi, rigore e integrità nell'amministrazione e nella destinazione delle risorse pubbliche. Nel distribuire le risorse, la finanza pubblica deve seguire i principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della valorizzazione dei talenti, e prestare grande attenzione a sostenere le famiglie, destinando a tal fine un'adeguata quantità di risorse. È con questa attenzione al bene comune che si è modulata la nostra azione legislativa, innanzi tutto in merito alle semplificazioni. Chi va in giro a incontrare "l'Italia che produce", le imprese, gli artigiani, i commercianti, i piccoli professionisti, il popolo delle partite IVA, ma anche i lavoratori dipendenti alle prese con la burocrazia,

miliardi. Le semplificazioni nel rapporto tra piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani e fisco, allora, sono state il nostro obiettivo principale: rispondono a tale obiettivo l'eliminazione delle *blacklist*, la sospensione degli accertamenti di agosto, l'accorpamento del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, la possibilità di pagare l'F24 in forma cartacea anche per gli importi superiori ai 1000 euro, il bollo virtuale sugli assegni circolari, le semplificazioni per gli enti e le organizzazioni iscritte negli enti beneficiari

anche per chi opta per la fatturazione elettronica, al fine di migliorare il sistema di comunicazione dell'IVA. E poi - e di questo andiamo particolarmente orgogliosi - il superamento degli studi di settore, sostituito con indici di fedeltà fiscale a cui sono legati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili anche in termini di esclusione o riduzione di termini per gli accertamenti al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari. Adottando questi indici cesseranno, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli odiati studi di settore. In poche parole i contribuenti più affidabili non avranno controlli e avranno rimborsi più ampi. Se le semplificazioni servono per predisporre al meglio il contribuente a soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole della riscossione significa che anche lo Stato deve fare la sua parte. Non ci sarà più Equitalia, si crea un nuovo ente pubblico economico che sarà ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, ma sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di 8.000 - con il loro grande bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. II nuovo ente di riscossione che nascerà nei prossimi mesi dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti lo statuto del contribuente, che riveda il sistema degli aggi e che si ispiri ai principi di cooperazione e di leale collaborazione. Potremo davvero aspirare ad avere un fisco non più inutilmente vessatorio e burocratico, ma più leale, più chiaro, più vicino alle esigenze dei contribuenti in difficoltà. Un fisco che valorizzi la sincera disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere con l'erario, ma nel contempo un fisco sempre più severo e intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada sbagliata di sottrarsi al proprio dovere tributario. Tutto questo è meglio ricordarlo in una cornice che, anno dopo anno, va svelando la sua concretezza e l'autenticità dell'impegno politico che la sta realizzando. Mi riferisco alla costante diminuzione della pressione fiscale dal 2014 al 2017, uno dei punti più qualificanti di questo Governo ed una novità assoluta per la politica italiana. Dopo la riduzione dell'IRAP, l'intervento sul reddito di lavoro subordinato, poi quello sulla prima casa e sull'IMU in agricoltura, per il prossimo anno il taglio dell'IRES con tre punti e mezzo in meno di aliquota, poi l'esenzione IRPEF ancora in agricoltura e quindi l'istituzione dell'IRI in favore di artigiani e di piccoli imprenditori.

l'annuncio della rottamazione delle cartelle e finalmente dell'abolizione di Equitalia. Eravamo tutti contenti; era stata finalmente accolta una richiesta del Movimento 5 Stelle, ma poi, quando si va a leggere il provvedimento, all'articolo 1,

"al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»" che "subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo Equitalia".

ogni anno intercorrerà un accordo tra MEF e direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà gli obiettivi quantitativi, l'ammontare delle entrate e la razionalizzazione delle risorse. Perché?

bastonati, anziché andare a recuperare l'evasione fiscale soprattutto delle grandi e grandissime imprese, delle banche e delle assicurazioni che spesso vengono lasciate libere di operare a danno di quei contribuenti che in realtà le tasse le pagano eccome.

Tali dati ci dicono espressamente che questo provvedimento non è un aiuto ai contribuenti, ma è un condono fiscale bello e buono, che serve a fare cassa per le mancette varie inserite nella legge di bilancio (non soltanto in questa, ma anche in quelle passate) e

fatto un'esposizione su come sono composte le cartelle non riscosse: il 3 per cento sono cartelle da 1 a 1.000 euro, cento da 1.000 a 5.000 euro, il 6 per cento da 5.000 a 10.000 euro. Questo sta a significare che i piccoli pagano, perché solo il 3 per cento delle cartelle che arrivano fino a 1.000 euro non sono pagate. Il grosso delle cartelle non riscosse sta nel 53 per cento che supera i 100.000 euro. Ma la questione fondante è che in questo 53 per cento la stragrande maggioranza è quella che va ben oltre i 100.000 euro, cioè che va sui milioni di euro, e che adesso potrà Ora, in un confronto televisivo con il vice ministro Zanetti ho fatto presenti queste criticità ed anche che quanto si va dicendo in giro a proposito dell'aggio non c'è in questo provvedimento, cioè l'aggio ci sarà ancora; lui invece mi ha risposto che verrà progressivamente eliminato. Dove sta, vice ministro Casero, la norma in cui si dice che progressivamente verrà eliminato l'aggio? Avete mentito per l'ennesima volta a quei poveri contribuenti che vorrebbero stare in regola, ma che non ce la possono fare, perché un sistema vessatorio, in questo momento di crisi, non può essere sostenuto. Non c'è scritto da alcuna parte, quindi per l'ennesima volta state mentendo. Lo stesso vale per quanto Non è che noi non vogliamo andare a cercare chi evade, però l'Agenzia delle entrate su questo punto è ancora in ritardo nel verificare tutte le dichiarazioni annuali Quindi mi chiedo, adesso che sarà travolta da queste dichiarazioni come farà a controllare e a velocizzare il controllo stesso. Ma qui si tratta sempre di imprese che hanno dichiarato e che non sono in grado di pagare. Voi dovete andare a cercare chi non dichiara e non fare, come avete fatto ancora in questo provvedimento, un nuovo condono per chi porta i capitali all'estero. Voglio capire: perché il *premier* Renzi andava in televisione, quando è stata fatta la prima *voluntary* *disclosure*, dicendo

Poi non diciamo che quei soldi torneranno in Italia per essere investiti, perché questa è un'altra megachiacchiera. Infatti quei soldi, che sono stati ripuliti, stanno rimanendo rimanendo all'estero e non stanno affatto ritornando qui per fare nuovi investimenti. Tra l'altro, le nuove normative, anziché semplificare (come è stato sempre sostenuto da questo Governo), stanno complicando; secondo la

100 euro per un anno! E gli aggiornamenti? E il pagamento del commercialista? 100 euro all'anno per un aggravio così sostanziale di tutta la normativa: ma vi

Vi abbiamo presentato emendamenti che sarebbero stati di buonsenso e presenteremo a breve anche un disegno di legge, mio e della senatrice Bottici, in cui chiediamo che, all'atto dell'avviso bonario, con una sanzione ridotta del 10 per cento, il contribuente possa pagare fino a 120 rate, senza passare dall'usuraio di turno, che in questo caso, anziché Equitalia si chiama Agenzia delle entrate riscossione. È questo il punto fondamentale.

XVII)*. Gentile Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Vice Ministro, rappresentanti del Governo, il decreto al nostro esame è un provvedimento che modifica una rilevante parte della normativa tributaria, per cui non si comprende l'uso del decreto-legge che, per l'occasione (come purtroppo in altre precedenti), ha beneficato coloro che ritengono il sistema bicamerale l'intralcio principe per la celere approvazione delle leggi, cioè un fattivo intervento del Senato. Il decreto in esame, pervenuto dalla Camera il 16 novembre 2016, deve essere convertito necessariamente entro il giorno 24 del corrente mese, perché le sue entrate sono di sostanziale supporto alla legge di stabilità

Inoltre, data l'urgenza del Governo, le Commissioni 5ª e 6ª non hanno potuto vagliare compiutamente gli emendamenti proposti, con l'ulteriore effetto che il provvedimento è privo di relatore. Peraltro alcuni degli emendamenti proposti - per grazia ricevuta - sono stati convertiti in ordini del giorno, la cui valenza è però a tutti nota. Data l'ampiezza degli argomenti trattati, mi limiterò a commentarne solo alcuni e, precisamente, l'articolo 6, relativo alla rottamazione delle cartelle. È un provvedimento di per sé positivo, anche in considerazione dell'ammontare degli insoluti, quasi inesigibili, presso gli esattori. Tuttavia esso non compendia tutte le necessarie fattispecie. Perché si rottamano solo le poste già affidate ai concessionari per la riscossione e si tralasciano quelle originate da atti pienamente dispositivi e, e, quindi, cogenti, ma non ancora affidate all'ente preposto alla riscossione? E ancora: quale differenza esiste tra una cartella esattoriale emessa da Equitalia, relativa alla sola sanzione tributaria, senza quindi debenza di alcuna imposta, e l'atto emanato da un ente con cui viene irrogata una sanzione per aver imbrattato un muro o affisso il manifesto «Vota Antonio» al di fuori degli spazi delimitati? Nessuna. Non soccorre alla bisogna l'articolo 6-*ter*, di nuova introduzione, anche perché non immediatamente operativo e comunque limitato alle sole poste di natura tributaria e previdenziale per la richiamata valenza del comma 10 dell'articolo 6, in evidente contrasto con la previsione del primo comma del detto articolo 6-*ter* secondo il quale sono ricomprese nella definizione agevolata le entrate anche tributarie e quindi tutte le entrate (le tributarie sono un "di cui"). Deve poi essere consentito al contribuente che abbia prodotto istanza di rottamazione di poter revocare tale istanza una volta che abbia preso visione del *quantum* della rottamazione comunicatagli dall'esattore, condizione assolutamente opportuna e necessaria per i ruoli per cui è in essere un contenzioso. l'articolo 4 e le norme per il recupero dell'evasione, tali disposizioni, di complessa natura, vanno poste in relazione stretta con l'articolo 7-*bis*, che disciplina la semplificazione degli adempimenti. Si aboliranno gli studi di settore una volta istituiti, con apposito decreto, gli indici sintetici di affidabilità: affidabilità: "apposito decreto" di cui non conosciamo compiutamente i termini. Tali studi di settore, peraltro, secondo quanto rilevato dalla stessa amministrazione finanziaria, non hanno punto contribuito all'emersione del sommerso e per di più sono stati raggiunti più volte dagli strali della Corte di cassazione che, giustamente, ne ha ridimensionato la valenza ai fini accertativi. Ma l'articolo 4, a fronte dell'abolizione dell'obbligo del cosiddetto "spesometro", che ha cadenza annuale, istituisce *ex novo* i seguenti nuovi obblighi a carico dei soggetti IVA: comunicazione telematica dei dati, tutti, delle fatture emesse e ricevute, vale a dire, mi si consenta, uno "spesometro" trimestrale; l'obbligo di comunicare, sempre telematicamente, i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali, secondo le modalità e con le indicazioni previste dal decreto IVA.

A fronte di tali onerosi adempimenti, il Governo ha segnalato che non esistono costi o misure aggiuntive, in quanto tutte le operazioni verranno effettuate automaticamente dai computer Qui non può sfuggire, però, che il contribuente dovrà comunque preparare quattro trasmissioni e che, ove lo stesso non sia in grado di formare il necessario *file* di trasmissione, dovrà affidarsi, come sempre, agli esperti del settore con quadruplicazione del costo. Se si considera, poi, che l'amministrazione finanziaria, ad oggi, sta vagliando le dichiarazioni IVA dell'anno 2014, ci si domanda quando verrà esaminata questa nuova mole di dati. Il dubbio è che si tratti di adempimenti non solo gravosi a dismisura, ma che ben poco contribuiranno al recupero dell'evasione. Un'ultima notazione: visto l'impegno del Governo a proporre nuove norme fiscali o a modificare il testo di quelle già esistenti, perché, finalmente, non si è posto termine al pasticcio della determinazione della "stabile organizzazione" per i professionisti ed i piccoli imprenditori ai fini dell'applicazione dell'IRAP? Un problema che attaglia decine di migliaia di contribuenti, in essere da più anni malgrado le ripetute indicazioni della suprema Corte di cassazione, rimaste però quasi del tutto inascoltate. Problema che ha prodotto un contenzioso stimato in migliaia di ricorsi alle competenti commissioni tributarie. Per tutti i motivi di cui innanzi, annuncio il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

il disegno di questo decreto-legge, correlato alla legge di bilancio 2017, è incentrato essenzialmente sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, Equitalia che viene annessa all'Agenzia delle entrate, la *voluntary disclosure* *bis*, la riforma degli studi di settore (sostituiti da indicatori di *compliance* fiscale) e numerose semplificazioni.

fondato sul reciproco affidamento, ciascuno nel rispettivo ruolo, uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela dell'interesse generale; nel contempo, si cerca di contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale.

dall'abolizione dei famigerati studi di settore, come già detto, alla modifica dei termini per gli adempimenti e versamenti di imposta; dalla sospensione dei termini nel mese di agosto alla dichiarazione integrativa in favore del contribuente; dalla semplificazione del regime della cedolare secca sugli immobili a quella sui rimborsi IVA e così via, con molte altre, attese da tanto Il decreto-legge interviene, inoltre, sulla riscossione, che è senz'altro il versante più delicato nel rapporto tra contribuente e fisco. Se le semplificazioni dovrebbero servire per mettere nelle migliori condizioni possibili il contribuente nel soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole della riscossione significa che anche lo Stato fa la sua parte. All'inizio ci sarà il superamento di Equitalia, con la creazione di un nuovo ente pubblico economico che sarà soggetto strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di ottomila - con il loro grande bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. Il nuovo ente di riscossione, che nascerà nei prossimi mesi, dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti quello del contribuente, che riveda il sistema degli aggi e si ispiri ai principi di cooperazione, di leale collaborazione e di affidamento, presenti nella legge delega. L'atto aggiuntivo alla convenzione annuale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, dovrà prevedere la tipologia di comunicazioni e di informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori anche mediante l'istituzione di uno sportello telematico secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di individuare con certezza il debito originario. Se tutto questo sarà realizzato conformemente alla volontà legislativa, avremo acquisito un buon risultato anche se non risolutivo. Meglio essere chiari: per ridisegnare il punto di equilibrio nel delicato campo della riscossione dei tributi è necessario intervenire anche nel settore delle sanzioni amministrative. Le semplificazioni e le nuove regole di ingaggio nella riscossione soddisfano il primo obiettivo, ovvero la costruzione del nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Ma un fisco non può permettersi di non insistere nel perseguire tenacemente il contrasto all'evasione fiscale, obiettivo fondamentale per qualsiasi strategia riformatrice oltre che politica, entrambe incentrate sull'equità e redistribuzione. Il fisco deve dialogare con il contribuente nella fase dichiarativa, deve informarlo nella fase che precede l'accertamento, deve porre il contribuente nella condizione di aderire, di ravvedersi e di rateizzare, deve informarlo prima della riscossione, deve essere chiaro e puntuale nella formazione del ruolo e nella redazione della cartella di pagamento e deve dare la possibilità di rateizzare. Deve fare tutto questo ed altro, ma al termine del percorso deve essere inflessibile con chi intenzionalmente si sottrae all'obbligo tributario in spregio dell'articolo 53 della Costituzione. Questo è il significato dell'articolo 3 del decreto-legge che affina e potenzia i poteri del nuovo ente di riscossione. L'ambizione del disegno di legge delega dovrà continuare a seguire questa strada e allora potremo davvero aspirare ad avere un fisco non più burocratico, ma più leale, chiaro e vicino alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, che valorizzi la trasparente disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere con l'erario. Nel contempo, avremo un fisco sempre più severo e - lo ripeto - intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada di sottrarsi al proprio dovere tributario. Sul decreto-legge alla nostra attenzione si potrebbe dire ancora molto, visto che è parte integrante dell'intera manovra di bilancio per il 2017, ma mi fermo qui, in quanto credo di aver riassunto i principali aspetti contenuti nel provvedimento e le ragioni atte a motivare un voto di fiducia favorevole

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Ruvolo.

di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: | |

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. Ha la parola la senatrice Bottici per illustrare la richiesta. colleghi, la cooperativa agricola «Il Forteto», fondata nella metà degli anni Settanta nell'azienda agricola di Bovecchio, Comune a Barberino di Mugello, è stata considerata per molti anni una delle principali comunità toscane di recupero di minori disagiati.

A me fa effetto dover chiedere per l'ennesima volta che su questa vicenda non ci sia più un velo oscuro. Dal 2013, quando sono entrata in quest'Aula, mi sono presa carico di quelle voci, di quelle vittime e di tutti i soggetti coinvolti. Ve l'ho chiesto in mille modi. Ho chiesto a tutti i parlamentari toscani di mettere veramente la parola fine a questa lunga storia. Gli orrori perpetuati

si parla di violenze di gruppo, di una manipolazione delle menti avvenuta cercando di cambiare

difesa in quest'Aula, per mettere al suo posto la famiglia funzionale, una famiglia fatta di rapporti omosessuali. Erano proibiti i rapporti tra uomo e donna perché serviva una famiglia funzionale. Veniva proibito ai bambini di vedere i propri genitori, perché erano affidati a queste famiglie funzionali. Mettiamoci nei panni di chi ha subìto e di chi ancora oggi è costretto a lavorare in quella cooperativa con i propri carnefici. Questa cooperativa esiste in Toscana, in Italia, che dovrebbe essere un Paese civile e democratico che tutela i minori e i più deboli;

che alcuni parlamentari provenienti dal Consiglio regionale della Toscana ancora oggi vogliano mettere

e ci hanno spiegato che hanno cercato di capire, di far emergere, di trovare quale parte della politica fosse coinvolta, quale parte della politica fatto sì che queste cose potessero andare avanti. Non è coinvolta solo la politica perché i tribunali, nonostante ci fossero delle sentenze contro i fondatori della cooperativa, hanno continuato essendo ben consapevoli di ciò a cui li mandavano incontro. È allora nostro dovere e nostro diritto, in qualità di cittadini, sapere come sono andate le cose. chiedo pertanto un'altra volta, con il cuore in mano, di non ostacolare l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, perché sicuramente qualcuno si alzerà in quest'Aula a dire che ci sono già state due commissioni d'inchiesta regionali.

ho parlato con una delle prime vittime che ho conosciuto e gli ho detto che non so come andrà, ma sono sicura di aver cercato in tutti i modi di far aprire gli occhi a quest'Assemblea e se essa riterrà essa riterrà di volerli tenere chiusi per l'ennesima volta e di proteggere quel sistema Forteto, collegato a fondi europei e regionali e alle cooperative,

come dovranno dormire quelle vittime che fino ad oggi non ci sono riuscite, perché speravano che la politica in qualche modo le potesse aiutare.

io che per decenni (prima da giornalista e poi da politico) mi sono occupato della questione relativa alla cooperativa "Il Forteto", combattendola con ogni mezzo, anche con interrogazioni parlamentari che non hanno mai avuto risposta, non posso che associarmi insieme al mio Gruppo alla richiesta di dichiarazione d'urgenza appena pronunciata dalla senatrice Bottici. Si potrà dire, com'è stato fatto, se un Consiglio regionale chiede al Parlamento di istituire una Commissione d'inchiesta, non è detto che il Parlamento automaticamente debba attivare Commissioni d'inchiesta su varie questioni che attengono ai vari territori italiani; tuttavia quello della cooperativa «Il Forteto» è uno scandalo nazionale nazionale che ha vissuto di coperture e di omertà per decenni, inspiegabilmente devo dire. È stato un sistema di potere radicatissimo,

ebbe poi a dire che non ci fu una sola telefonata, ma una serie di telefonate di avvertimento perché non si pronunciasse nemmeno il nome «Forteto», in tanti anni di lavoro - e gli anni di lavoro giornalistico di Vespa sono davvero molti - non aveva mai ricevuto così tante pressioni e che solo allora aveva capito davvero la forza di questa Credo che il muro di gomma che c'è stato per più di trent'anni (dal 1977) debba essere finalmente spazzato via, quindi la richiesta di una Commissione parlamentare non è strumentale. Non è solo un atto dovuto, ma un impegno politico e soprattutto morale che non può essere eluso da questo Parlamento.

ci ha chiesto - questo è il punto - una Commissione parlamentare d'inchiesta (che ha poteri equiparabili all'autorità giudiziaria) per arrivare dove finora non si è potuto o non si è voluto arrivare, perché le zone d'ombra e i punti oscuri restano ancora molti. Quindi, bisogna assolutamente squarciare il velo di omertà e di menzogne

disagiati, finiti in mano a un gruppo di pedofili grazie all'incredibile distrazione dei tribunali per i minorenni, dei servizi sociosanitari, delle istituzioni tutte. Un sistema, al quale una parte della politica non è stata purtroppo estranea, che ha permesso ai fondatori del Forteto di calpestare la dignità e i diritti umani di decine di bambini, di schiavizzarli, di allontanarli dalla propria famiglia, di annientarli psicologicamente, di violentarli sistematicamente,

una comunità e poi un'associazione, una fondazione, una cooperativa, ma anche ai suoi vertici un'associazione per delinquere, come hanno certificato le sentenze della magistratura, anche queste arrivate con incredibile e colpevole ritardo. Dunque, ora è il momento che anche il Parlamento faccia la propria parte per mettere la parola fine a questa decennale vergogna italiana - non toscana, ma italiana per fare definitivamente giustizia. Termino il mio intervento ricordando che il caso è nazionale, perché siamo in presenza di persone condannate in via definitiva per violenza su minori nella stessa struttura cui lo cui lo Stato per decenni ha continuato ad affidare i bambini. Se questo non è uno scandalo nazionale su cui fare definitivamente luce, ditemi voi cos'è. Confermo pertanto il nostro voto favorevole alla dichiarazione di urgenza.

presentata dalla senatrice Bottici, e lo faremo perché pensiamo che sia un atto dovuto per una delle più brutte pagine che riguardano

venivano via dalle proprie famiglie, dove avevano subito abusi, povertà, difficoltà e disagio sociale. Quello che è successo

lo ha raccontato in parte anche il lavoro che sta facendo la magistratura, non ancora completo, ma tutto ancora da proseguire. Credo che proprio per la drammaticità di quei fatti e per la gravità

deve essere portato avanti con i poteri e gli strumenti che il Parlamento può mettere a disposizione, come quelli di una Commissione di inchiesta. Riportare

questo lavoro con senso di responsabilità, ma soprattutto per amore della verità. Lo dobbiamo ai tanti ragazzi che sono stati ospiti del Forteto e che con difficoltà, ancora oggi, raccontano cosa hanno vissuto e subito. Oggi, provano a uscire da quella situazione difficile di ulteriore disagio, anche grazie a progetti che la Regione Toscana, insieme ad alcune associazioni

il voto di oggi sia un atto dovuto che il Parlamento deve a una storia troppo a lungo silenziata e che ha bisogno invece della giusta verità. Per questo motivo voteremo a favore.

il Gruppo di Forza Italia sosterrà con molta forza la richiesta della senatrice Bottici, che ringrazio per avere

è intorno a quell'abominio di violenze su minori, bambini disabili, ai vari suicidi, stupri e alla rovina della vita delle vittime. vittime. Quella comunità ricevette un finanziamento, dal 1996 al 2010, di oltre 1,2 milioni di euro dalla Regione Toscana nonché fondi dalla Comunità europea. Si sperimentava omosessualità, pedofilia, zoofilia: tutto quello che era la negazione della natura, quasi come se regnasse un'anarchia morale. Si sarebbe potuto fermare tutto questo un anno dopo l'apertura, quando un magistrato arrestò il fondatore Roberto Fiesoli per violenza sessuale. Ma non servì. Venne scarcerato e ci fu una presa politica fortemente ideologica della comunità che lo sosteneva con l'affermazione che le denunce di violenza erano solo frutto di malelingue. Fiesoli si faceva chiamare il profeta. Riuscì - non si sa bene come, vista la scarsa credibilità che avrebbe dovuto avere - a organizzare - a organizzare conferenze. Antonio Di Pietro tenne persino una conferenza contro la pedofilia; passarono Livia Turco, Rosi Bindi, Fassino,

siffatta richiesta possa essere condivisa da tutta l'Assemblea. Dalla Commissione di inchiesta della Regione Toscana emerse che la prassi della comunità Il Forteto risultava essere l'abuso.

Signor Presidente, noi non ci opporremo alla richiesta della dichiarazione di urgenza e, quindi, voteremo a favore. E lo faremo consapevoli della complessità della vicenda

che difficilmente una nuova Commissione d'inchiesta sul piano strettamente delle sentenze e delle condanne potrà aggiungere molto. entriamo in una prassi nella quale tutte le vicende regionali finiscono per arrivare in Parlamento, con la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta nazionale è evidente che ci mettiamo su un terreno abbastanza complicato da gestire, ancor di più se si ritiene che quelle Commissioni debbono avere caratteri giudiziari che si sovrappongono e spesso contrastano con le attività che la magistratura ha già svolto. però di questioni che casomai vedremo nel momento in cui si affronterà il tema dell'esatto mandato che la Commissione d'inchiesta avrà. In questo momento voglio dire che, di fronte a una richiesta unanime del Parlamento, noi non ci tiriamo indietro, anche perché non c'è niente da nascondere sul piano né politico né personale e, quindi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore.

all'istituzione della Commissione d'inchiesta per le motivazioni che abbiamo ascoltato e che condividiamo, ma anche per le perplessità legate al

e bene le commissioni d'inchiesta regionali. Abbiamo ascoltato che due commissioni d'inchiesta della Regione Toscana hanno già lavorato

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, il termine residuo per la presentazione delle relazioni, previsto dall'articolo 44 del Regolamento, viene ridotto alla metà. Inoltre, in coerenza con precedenti decisioni assunte durante i recenti lavori di questa Assemblea, la Presidenza precisa che, qualora in seguito la Commissione competente provveda alla connessione della proposta con altri disegni di legge, il dimezzamento di tutti i termini di esame, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, si estenderà anche ad essi.

si restringe l'applicazione delle linee guida alla sola imperizia e si mantiene la punibilità per le altre due forme, la negligenza e l'imprudenza, anche se l'esercente la professione sanitaria si è astenuto nelle raccomandazioni di diligenza e prudenza contenute nelle stesse linee guida.

e 45527 del 2015). La formulazione attuale comprenderebbe pertanto una previsione peggiorativa rispetto la disciplina attuale e la sua interpretazione giurisprudenziale. Si ritiene inoltre che l'inciso «salvo la specificità del caso concreto» consenta al giudicante di valutare dette specificità senza che la stessa valutazione sia vincolata all'adeguatezza delle linee guida nel caso specifico.

il pubblico ministero rinvia direttamente al giudice che emette la sentenza. In coerenza con quanto stabilito dall'attuale rito del processo penale, chiedo che si passi attraverso l'udienza preliminare. Una situazione analoga si è presentata per il reato di diffamazione. Vi è stata una valutazione, fatta anche dal giudice delle leggi (con la sentenza n. 68 del 1991), che ha recuperato un diritto in capo al soggetto imputato di quel reato - mi riferisco al reato di diffamazione, che generalmente riguardava i giornalisti

ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibile per estraneità all'oggetto del disegno di legge l'emendamento

che sanciscono l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario nazionale di rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, immediatamente e direttamente per i fatti illeciti dei loro funzionari e dipendenti e, pertanto, dei danni dagli stessi causati al terzo paziente.

è una specifica che con il mio emendamento - a mio parere - vado a semplificare. Infatti, la specifica dice: «salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente», e quindi il giudice, nel determinare il danno, tiene conto della condotta dell'esercente. Credo Credo di poter semplificare la situazione che viene creata con questo inciso con una formulazione molto più diretta che riconduce tutto esclusivamente ai casi di dolo o di colpa grave. necessario per una maggiore chiarezza e per la comprensione di tutti, ma anche per una semplificazione che di questi tempi credo sia sempre importante.

Inserendo questo piccolissimo inciso - secondo il mio parere - si potrebbero meglio definire i contenuti della parola «contrattuale». infatti, che, se vi era stato un precedente rapporto tra medico e paziente, allora si incardina quella contrattuale, altrimenti resta in vigore quella extra contrattuale.

l'obbligo di rispettare le norme del codice della strada che grava su un automobilista, perché è questa, in pratica, la differenza della responsabilità *ex* articolo 1218 ed *ex* articolo 2043 del codice civile. Mi sono confrontato - e ringrazio per questo il relatore - anche rispetto alla giurisprudenza, immaginando, dalla prima lettura della norma, che potesse essere cambiata. Devo dire Devo dire che, facendo una ricerca, dopo la legge Balduzzi del 2012, vi sono state solamente quattro sentenze - due del tribunale di Milano, una di Varese e una di Torino - che seguono la tesi del del rapporto extra contrattuale del medico. Quattro sentenze su circa 6.000/8.000 rappresentano un numero davvero risibile.

nella quale fondamentalmente vengono stabilite le responsabilità contrattuali sia del medico che della struttura sanitaria, isolando quelle pochissime sentenze contrarie di merito che andavano nella direzione opposta e che ho citato prima. Con la sentenza n. 64440 del 2015, che tratta una vicenda di responsabilità professionale che vedeva convenuti la struttura sanitaria e il medico ginecologo nella fattispecie, che era dipendente della struttura sanitaria, struttura sanitaria, si è ribadito che il fatto illecito si innesta nell'inquadramento contrattualistico del contatto sociale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte.

ritenendo che questa locuzione, secondo l'intendimento di chi propone questo tipo di provvedimento, possa risolvere così il problema, ritiro l'emendamento che ho illustrato. E l'ho illustrato perché rimanga gli atti, in quanto ho il dubbio che, nonostante le buone intenzioni del legislatore, non è detto che raggiungiamo il risultato in sede giurisdizionale quando si verificheranno cause in materia.

visto che il senatore Cuomo ha illustrato in modo egregio il suo che è identico al mio. E, per le stesse motivazioni, lo ritiro.

senatori D'Ambrosio Lettieri come ben sanno il relatore e il Governo (come hanno potuto evidenziare in sede di dibattito in 12a Commissione), uno dei temi su cui si è registrata qualche criticità è proprio quello dell'azione del risarcimento. vi è una differenziazione delle norme fra i medici dipendenti, per i quali l'azione di risarcimento è riferita ai cinque anni, e i liberi professionisti, per Relativamente a questo, che è uno dei temi più delicati affrontato, anche in modo assolutamente coerente con l'esigenza, l'esigenza, sarebbe opportuno prevedere un limite temporale all'azione del risarcimento, che fisso in due anni; termine che dovrebbe decorrere dall'esecuzione dell'atto medico e non dalla mera presa di coscienza del danno.

7.210 chiedo di inserire, alla fine del comma 4, «non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138». Come ho già detto anche in sede di discussione generale, ritengo che bisogna rimuovere questo limite per affidarci all'operato dei giudici, i quali meglio di noi sapranno, caso per caso, adeguare la liquidazione dei danni alle circostanze della vicenda giudiziaria giudiziaria di causa. Quel limite serve nella responsabilità civile auto, solo perché controbilanciato dal fatto che i premi assicurativi

riguarda l'intero impianto del risarcimento del danno e la struttura nella sua interezza. Sinceramente non ritengo giusto il motivo per cui dobbiamo ridimensionare i danni a favore della vittima, facendo implicitamente un danno alle potenziali vittime e favorendo - invece - le strutture sanitarie o le assicurazioni laddove dovessero contrarre polizza.

sull'ultima riflessione svolta dal senatore Cuomo. In realtà, il provvedimento nella sua organicità prevede il risarcimento dei danni provocati sia dai professionisti che dalle strutture in base a tabelle

Nel provvedimento c'è il riferimento specifico a detto aspetto e, quindi, tutto si svolgerà per la personalizzazione del danno, che è il tema caro al senatore Cuomo e - devo dire - a tutti, perché dà certezza

Il dubbio che è sorto ai colleghi Cuomo, Ranucci e ad altri sentori di parti politiche diverse impone a un legislatore corretto di tener conto del dubbio interpretativo che si è posto e di risolverlo attraverso la specificazione. un'espressione inutile, ma è preferibile rispetto al fatto di lasciarlo appeso di modo che non si sa se l'affidamento è compreso o no. Ciò determinerà un'interpretazione da parte del giudice

legislativa e diventa complicata anche la gestione di questo articolo così come proposto. Faccio quindi un semplice riassunto. La procedura conciliativa, nell'ambito della mediazione obbligatoria disciplinata dal decreto-legge del 2013 (che oltretutto segue una procedura del tutto analoga a quella disposta dall'articolo 8 del presente disegno di legge e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013), già si pone come condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione giudiziale e come strumento idoneo a stimolare le parti alla composizione stragiudiziale si ritiene che l'introduzione del nuovo strumento processuale, dato dal procedimento obbligatorio di cui all'articolo 698-*bis* del codice di procedura penale, sostanzialmente sovrapponendo la nuova procedura a quella preesistente, ponga inoltre problemi interpretativi di coordinamento proprio con le norme di detto decreto-legge n.

all'inizio dell'articolo per definire meglio le due alternative a cui il cittadino può fare riferimento, ma nel caso non ho alcuna difficoltà a convergere sottoscrivendo l'emendamento 8.206 del collega D'Ambrosio Lettieri, che ritengo sostanzialmente simile al mio. Ribadisco al Governo e al relatore

di verificare, in relazione ai due emendamenti se la tecnica legislativa e la valutazione lessicale degli emendamenti, possa consentire di intervenire al comma 1 anziché al comma 2. Questa è una vicenda squisitamente tecnica, perché nella sostanza non cambierebbe nulla, atteso che la mediazione sarebbe

che all'articolo 5, comma 1-*bis*, introduce l'istituto della mediazione che nell'ambito della responsabilità medica e sanitaria in generale ha avuto

ha la finalità di allontanare dal processo, e quindi dall'aula del tribunale, un contenzioso avvicinandolo a una mediazione che può,

tutti gli aspetti che concorrono a sostenere l'esatto opposto, ed in tal senso sono formulati i miei emendamenti: meno costi, effetto deflattivo sul contenzioso nelle aule dei tribunali e io credo anche una efficacia maggiore nel conseguimento del risultato che le parti possono conseguire in una conciliazione che la mediazione agevola.

che tecnicamente si pone meglio perché contestualmente sopprime quel periodo che vieta la mediazione, quindi da questo punto di vista funziona meglio; ciò tenuto conto che non abbiamo nulla da aggiungere sulla conciliazione, perché finalità e procedure fanno già parte dell'ordinamento vigente.

La materia era molto tecnica e molto perimetrata su competenze rilevanti soprattutto del Ministero della giustizia. Ovviamente il nostro lavoro in Commissione è stato in perfetta e totale

apprezzate le circostanze, L'Assemblea tornerà a riunirsi sempre martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.